oggi la politica italiana ha perduto una delle protagoniste di una stagione ricca e controversa, quella delle conquiste femminili in termini di diritti e libertà. Oggi ci ha lasciato Alma Cappiello, colei che, in quegli anni, illuminava con il suo solare sorriso il percorso, a volte accidentato, del ruolo delle donne in politica e nelle istituzioni. Tra gli anni Ottanta e il 1995, le donne italiane vivono una stagione politica e istituzionale assai interessante: dalla creazione degli organismi di parità alle azioni positive nel lavoro dipendente, nel lavoro autonomo e nella politica. Tutto ciò nella cornice europea e delle Conferenze dell'ONU di Nairobi prima e di Pechino poi. Temi come la giustizia sociale nella visione dei meriti e dei bisogni di un moderno *Welfare* *State*, la famiglia, la procreazione assistita, la riforma dell'affido e delle adozioni e, soprattutto, la realizzazione della democrazia paritaria nella politica, nel lavoro, nell'economia e nella finanza erano il pane quotidiano di Alma Cappiello. Nelle istituzioni è consigliere comunale a Milano nel 1985, deputata, responsabile della Commissione nazionale per la parità presso la Presidenza del Consiglio e, soprattutto, dirigente nazionale del Partito socialista italiano, di cui diventò la responsabile femminile dopo la senatrice Elena Marinucci. Ella chiude un filo di perle lungo cento anni di socialismo riformista, che ha visto brillare figure fulgide come Anna Kuliscioff, teorica del riformismo e madre della prima legge di tutela della maternità, come Argentina Altobelli, prima segretaria del sindacato dei braccianti (allora il più potente), come Anna Maria Mozzoni, fondatrice dei primi asili nido sui luoghi di lavoro in quella Milano culla del riformismo, e come Lina Merlin, che mise fine al commercio di carne umana legalizzata nelle case chiuse. Cento anni di socialismo conclusi nell'ultima responsabile femminile, Alma Cappiello, che dovette penare molti anni, insieme con tante di noi, per vedere approvata dal Parlamento italiano la legge contro la violenza sessuale. Quel soffitto di cristallo, che anche lei combatteva, non è ancora infranto e non tutti i diritti di cittadinanza, ancorché scritti sulla carta, si sono ancora compiutamente realizzati. non l'ha vinta l'ingiustizia politica di veder finire con lei la storia del Partito socialista italiano. L'ha vinta invece un male tremendo che l'ha piegata fino alla fino alla morte, ma fino all'ultimo è rimasta vicino alle lotte anche moderne delle donne italiane per ribadire, conquistare e riconquistare pezzi di libertà. Oggi certamente il suo pensiero era rivolto, così come in tante di noi, a quelle donne e a quelle sorelle che girano per le nostre strade con il capo coperto in virtù di una legge assurda che qualcuno chiama Corano, ma che in realtà è solo è solo un arcaico e quanto mai ottuso modo di intendere le diversità tra uomini e donne. Il nostro pensiero va ad Alma Cappiello e alle contaminazioni che, insieme con molte parlamentari e colleghe del suo tempo, è riuscita a svolgere nelle diverse aree politiche. Le senatrice e i senatori di Forza Italia oggi la piangono.

per portare a conoscenza la Presidenza e i colleghi di una questione che ha riguardato oggi la Commissione affari costituzionali. Si tratta di una questione regolamentare, che ritengo di estrema delicatezza, senza voler naturalmente aprire polemiche, perché anche il Presidente della Commissione non ha forse inteso la portata - diciamo - innovativa e rivoluzionaria di alcune norme che ha ritenuto di ricavare dal Regolamento del Senato, applicandole in Commissione, in materia di parere che la 1a Commissione deve

per cui anche il voto diventa una specie di operazione al cardiopalmo perché non si sa mai se vi è un senatore in più o meno rispetto alle maggioranze che sono presenti *per* *tabulas*. Il presidente Bianco - utilizzando una norma regolamentare scritta per l'Aula e considerando, giustamente per questo aspetto, questo aspetto, che il voto della Commissione sui presupposti rappresenti una condizione procedimentale del decreto-legge e quindi dovesse avere una corsia speciale - ha ritenuto, senza verificare nemmeno i tempi necessari per lo svolgimento completo della discussione e per il voto, di attribuire dieci minuti a ogni Gruppo Gruppo per la discussione generale, naturalmente innovando profondamente la prassi parlamentare. Si tratta di un'innovazione che non trova alcun collegamento, alcun riferimento testuale nei lavori di Commissione.

il provvedimento della Presidenza: per noi non ha alcun valore in quanto si tratta di una decisione che non trova riscontro nel Regolamento né nei precedenti. Vorrei, però, che la Presidenza si facesse carico di un chiarimento su questo punto, invitando tutte le forze politiche a lavorare, senza venir meno alle prerogative di ciascuno, con

per eventuali prese di posizione sulla questione da lei sollevata. Come lei sa, il Regolamento prevede che la 1a Commissione ha cinque giorni di tempo per esprimere il proprio parere. Nell'ambito del Regolamento, informeremo

Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola e voglio porre alla sua attenzione ed a quella dei colleghi un fatto che si è verificato su Internet e che mi è stato segnalato da associazioni di genitori di bambini Down*.* Risultano presenti su Internet due siti, dove si evince una classe di ragazzi italiani, all'interno della quale vi è un ragazzino Down, schernito, deriso e maltrattato verbalmente dagli altri compagni. Vorrei segnalare a lei e all'Assemblea questo fatto affinché vengano adottati tutti i provvedimenti utili (perché dal sito non è possibile risalire alla paternità

danneggiano sicuramente i ragazzi Down e le loro famiglie, ma credo anche la dignità di tutti noi. Voglio esprimere un profondo rammarico e dissenso per quanto è avvenuto e mi auguro che al più presto

Presidente, dal momento che è intervenuto il senatore Pastore adducendo che vi erano stati oggi momenti di difficoltà e forse di irregolarità nei lavori della Commissione affari costituzionali e dal momento che lei giustamente si è riservato di rappresentare questa situazione alla Presidenza,

a verbale che non condivido affatto l'impostazione del collega Pastore. Non c'è stata alcuna compressione, alcuna irregolarità, assolutamente, nei lavori di oggi in Commissione. Non c'è stata neanche alcuna prevaricazione da parte del presidente Bianco che, a mio modo di vedere, ha correttamente interpretato il Regolamento. Tant'è vero, i fatti alla fine parlano, che non siamo nemmeno arrivati al voto. C'è stata solo un'ampia discussione e si voterà domani. Quindi, non si può dire che si è cercato di affrettare la decisione della Commissione e di comprimere i diritti di ciascun senatore o delle parti politiche. Vorrei segnalare che quel che sta davvero accadendo è che, essendo i numeri in Commissione ovviamente quelli che riflettono l'equilibrio complessivo tra le forze politiche nell'intero Senato, si determinano situazioni in cui l'opposizione, del tutto legittimamente, voglio dirlo in chiaro, cerca di creare difficoltà alla maggioranza e di approfittare del momento più favorevole, di qualche occasionale assenza, e cose di questo genere. Ribadisco che è un comportamento del tutto legittimo, che però si sta traducendo in uno spezzettamento delle decisioni della Commissione, nel tentativo di moltiplicare artificiosamente le occasioni di voto, perché ogni voto dal punto di vista dell'opposizione diventa una possibile per la maggioranza. Quindi, soprattutto sui presupposti dei decreti-legge, voti nei quali si determina il rischio potenziale della caduta del decreto, stiamo andando

tecnicamente ineccepibile dal punto di vista di chi lo propone, ma è ovvio che pone una questione di complessiva disciplina dei lavori della Commissione, perché non si può leggere mai il Regolamento nel senso del blocco dell'istituzione o della determinazione dell'impossibilità dell'istituzione a decidere. E questo vale, sia per l'Aula sia per le Commissioni. Il presidente Bianco oggi ha fatto richiamo, come

Fazio, Sodano, Battaglia Antonio, Libè, e registra quindi un'ampia convergenza del Senato in occasione della Conferenza internazionale delle Nazioni Unite di Nairobi,

La Commissione europea, in occasione di questa Conferenza, ha inviato una comunicazione nella quale si legge che i dieci anni più caldi mai registrati sono concentrati dal 1991 in poi che le concentrazioni di gas serra sono le più elevate degli ultimi 450.000 anni. Stiamo quindi parlando di un tema cruciale per il presente e per il futuro dell'umanità.

poiché dal 1990 al 2003 tali emissioni sono aumentate del 18 per cento, la Commissione europea indica come obiettivo attuale un'effettiva riduzione del 33 per cento. Quindi, è un grandissimo impegno che viene proposto.

Gli incrementi più consistenti hanno riguardato il settore dei trasporti, più 27,5 per cento, e quello della produzione di energia termoelettrica (più 17

Per l'Italia è molto importante collegare l'impegno di Kyoto con la riduzione del consumo di combustibili fossili. L'Italia ne ha consumati nel 2005 185,9 milioni di tonnellate, per il 91 per e la bolletta energetica ci è costata nel 2005 36,5 miliardi di euro. Si tratta quindi di fare dell'attuazione del Protocollo di Kyoto un'occasione per ridurre la dipendenza dai combustibili in particolare nei settori a più alto consumo, nel settore dei trasporti ma anche in quello dell'energia elettrica, degli usi civili e del terziario, con misure di efficienza energetica, con lo sviluppo del cabotaggio, del trasporto su ferro e collettivo, con maggiore consistente impegno per la produzione e l'uso di fonti rinnovabili pulite per generare energia elettrica, calore, carburanti, con possibili ricadute positive tecnologiche produttive e anche occupazionali. La mozione impegna il Governo ad operare per ampliare la partecipazione a iniziative per affrontare il cambiamento climatico. Poiché sei Paesi (Stati Uniti, Canada, Russia, Giappone, Cina e India), insieme all'Unione Europea, Europea, producono il 75 per cento delle emissioni mondiali di gas serra, la mozione invita: a sostenere gli sforzi tesi ad attivare e a trovare un'intesa fra questi grandi Paesi emettitori, una sorta di G7 per il clima; a sostenere la ricerca, il cambiamento tecnologico e l'economia della conoscenza; ad attuare il Protocollo di Kyoto come occasione per ridurre la dipendenza del combustibile fossile e la fattura delle importazioni energetiche del Paese; ad aggiornare la delibera del CIPE n. 123 del 2002 e il relativo Piano nazionale di riduzione dell'emissioni, in modo da far fronte alla crescente distanza (lo ripeto, 97,7 milioni di tonnellate di CO2) dall'obiettivo di Kyoto; a integrare il Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas serra in un programma nazionale energetico-ambientale, concordato con le Regioni e anche con obiettivi regionali

a rafforzare la ricerca ed il supporto tecnico alla diffusione delle politiche e delle misure che concorrono alla riduzione delle emissioni di gas serra; a prestare grande attenzione al settore dei trasporti, della mobilità e della logistica; a fare dell'efficienza e del risparmio energetico un'effettiva priorità; a promuovere con maggiore efficacia lo sviluppo di tutte le fonti energetiche rinnovabili (idriche, geotermiche, eoliche, solari, biomasse) per la produzione di energia elettrica di calore e di carburanti, superando i certificati verdi e l'incentivazione delle fonti non rinnovabili assimilate con un sistema incentivante differenziato per fonte, senza tetti, accessibile, certo e di lunga durata, assicurando il collegamento con le reti di distribuzione e procedure di localizzazione e di autorizzazione più semplici; a sostenere, in rapporto con le piccole e medie imprese, la piccola generazione distribuita, di energia elettrica e di calore, che consente maggiore efficienza e più alti rendimenti; a sostenere lo sviluppo dei distretti agro-energetici modo che l'agricoltura possa valorizzare sia le risorse locali, sia nuove produzioni; a sostenere la ricerca e la sperimentazione della cattura e del sequestro sicuro della CO2, così come dello sviluppo dell'idrogeno.

Presidente, nel 2002, un anno dopo il successo elettorale del centro-destra, venne ratificato il Protocollo di Kyoto. Va sottolineato che i Governi di centro-sinistra,

dei gas serra in Italia avevano registrato un balzo in avanti, come pure la crescita di energia da idrocarburi altamente inquinante.

Non solo: nei cinque anni di Governo Berlusconi è unanimemente riconosciuto che l'Italia ha registrato i maggiori *standard* di efficienza energetica, che l'apparato produttivo del Paese si è dotato di processi innovativi tali da permettere a questo Paese, all'Italia, di registrare in Europa i maggiori *standard* di efficienza energetica.

Ora il Paese si trova di fronte alla necessità di ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra del 6,5 rispetto ai livelli del 1990 e deve realizzare questo impegno tra il 2008 e il 2012.

e quella liberal-democratica della condivisione e del partenariato. Il Governo Berlusconi ha seguito questa linea coinvolgendo le imprese nazionali in azioni che potessero diventare economicamente vantaggiose;

Va poi sfatata qualche leggenda metropolitana. Per esempio, qualcuno sostiene che il Canada, un Paese governato fino a poco tempo fa

Per quanto riguarda la produzione di inquinamento atmosferico *pro* *capite*, il Canada inquina molto più degli Stati Uniti. In realtà, Presidente - tanto per riferirci a qualcosa di concreto e di reale - in Francia, per esempio, i bovini emettono gas serra tre volte superiori alle raffinerie di petrolio, ben 14, presenti nel Paese. Quindi, in realtà, il gas serra non è prodotto soltanto dall'inquinamento atmosferico dovuto ai motorini o alle auto, ma anche...

Noi con il Governo Berlusconi tentammo di risolverlo e l'avviammo a soluzione con i permessi di emissione, con i meccanismi flessibili, con quella che era l'attuazione congiunta del Protocollo di Kyoto; tutti sistemi che permettevano anche forme di finanziamento allo sviluppo sostenibile dei Paesi del Terzo mondo. Questa è una linea da seguire ed è una linea sulla quale noi chiediamo al Governo di impegnarsi.

ringraziamo il Ministro per la sensibilità mostrata a discutere di questo importante argomento oggi nell'Aula del Senato. II rapporto 2006, presentato in questi giorni dal WWF, lancia l'ennesimo allarme per il futuro del pianeta: se continua l'attuale ritmo di consumo di acqua, suolo, risorse forestali e specie animali, nel 2050 saranno necessari 2 pianeti per il sostentamento della popolazione mondiale in crescita. Consumiamo le risorse più velocemente di quanto la terra sia capace di riprodurle e immettiamo scarti che il pianeta non riesce più a metabolizzare. Il cambiamento climatico tocca tutti noi. Adesso è una nostra responsabilità primaria fermarne le disastrose conseguenze e i dati scientifici attestano la gravità della situazione. La Royal Society, il 4 settembre scorso, ha denunciato pubblicamente la pratica della Exxon di creare e sostenere associazioni ambientaliste con il solo scopo di alimentare il dubbio sulla realtà e sulla portata del cambiamento climatico. La ExxonMobil, nel solo 2005, ha speso ben 2,9 milioni di dollari per finanziare una quarantina di organizzazioni al fine di fornire informazioni distorte sui dati scientifici relativi al cambiamento climatico, di negare gli evidenti effetti delle emissioni di gas serra, di sovrastimare l'incertezza e il dubbio. Così come non è sulla capacità di adattamento dell'umanità che bisogna puntare per affrontare seriamente questo problema globale. L'insicurezza climatica è direttamente collegata alla dipendenza da combustibili fossili ed è sentita sia nei Paesi ricchi che in quelli poveri: dai villaggi costieri del Pacifico meridionale che si spostano verso l'entroterra per evitare l'avanzata del mare, alle mortali ondate di calore che colpiscono l'Europa, agli uragani distruttivi che colpiscono gli Stati Uniti d'America. Contrastare gli effetti climatici è una necessità e noi auspichiamo che il Governo Prodi, così come già nel programma dell'Unione, si è impegnato a raggiungere almeno l'80 per cento degli obiettivi di riduzione attraverso l'incremento dell'efficienza delle fonti rinnovabili e, tuttavia, in questo crediamo che bisogna fare di più. Il 13 ottobre scorso, un importante impegno del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente hanno raggiunto un accordo per il Piano nazionale delle emissioni. Ancora poco, bisogna fare di più e noi speriamo che la Conferenza di Nairobi possa rappresentare l'impegno concreto del Ministro e del Governo perché si volti definitivamente pagina su questo tema. È obbligatorio non perdere di vista la dimensione globale della problematica e tenere i Paesi in via di sviluppo in debita considerazione nel futuro regime internazionale per la lotta al cambiamento climatico. E questo è uno dei punti più sensibili della nostra mozione...

Signor Presidente, colleghi senatori, la prossima Conferenza di Nairobi tra le parti firmatarie del Protocollo di Kyoto impone un'analisi attenta e matura della posizione e dei provvedimenti adottati da tutti i Paesi. La questione ambiente è problema grosso, di quelli che accomunano i popoli. Certo, il ritiro dei ghiacciai, l'innalzamento del livello del mare e delle temperature, la siccità e le alluvioni rappresentano emergenze da affrontare con piani nazionali ed internazionali *ad hoc*. Non basta firmare un accordo tra Stati per sentirsi appagati moralmente: la coscienza al sicuro esige concretezza e operatività. Va bene la poca tolleranza verso chi non rispetta i limiti delle emissioni; va bene rifiutare sanatorie; va bene il segnale di svolta dato con l'ultimo accordo tra i ministri Pecoraro Scanio e Bersani per tener fede agli impegni di riduzione delle emissioni dei gas responsabili dell'effetto serra e del riscaldamento del pianeta. però, deve seguire l'attuazione concreta dell'impegno del Governo come occasione di rivincita del pianeta sulle manovre invasive di sfruttamento artificiale e sull'abuso dell'umanità industrializzata e consumistica. Il nostro Paese, ancorché piccolo rispetto ad altri, è una delle potenze industriali mondiali, che deve fungere da esempio. Sono d'accordo ad impegnare il Governo, come richiesto dalla mozione, ad attivarsi in azioni che si concretizzino in opportunità di sviluppo sostenibile e di riconversione ecologica dell'economia, in incentivo alla produzione agricola contro l'abbandono dei campi, in opportunità di sviluppo agro-energetico. Proprio il campo dell'agro-energetico, ponendo in sinergia la ricerca e l'innovazione tecnologica con lo sviluppo dell'agricoltura e determinando la riduzione delle emissioni gassose, rappresenterebbe una risposta alle problematiche ambientali connesse all'applicazione del Protocollo di Kyoto. Tra l'altro, il rispetto dei parametri di emissione verrebbe agevolato da una politica di promozione delle energie alternative e rinnovabili: vento, acqua, sole e biomasse, come risorse energetiche, rappresentano una risposta alla problematica dei gas inquinanti che il Governo non può sottovalutare. Onorevoli senatori, gli studiosi prevedono un innalzamento delle temperature da due a sei gradi, con estati da record, dati che richiedono urgenza e concretezza. Perciò, è importante rispettare i traguardi di Kyoto, che sono progettazione orientata al lungo periodo. Ebbene, la XII Conferenza mondiale sul clima che si terrà a Nairobi dovrebbe stabilire proprio un calendario di lavoro, nel quale si fisseranno gli obiettivi per il periodo successivo al 2012. Il nostro Paese non può che impegnarsi al rispetto massimo del piano, visto che i risultati degli obblighi assunti (ridurre le emissioni dei gas serra del 6,5 per cento, parametro previsto dal 2008 al 2012)

questa volta alle parole dovranno seguire i fatti, le azioni ed i provvedimenti, perché non possiamo più accontentarci di promesse o di tentativi improvvisati. Se non rispettiamo operativamente le disposizioni limitative dei patti, non possiamo alzare la voce contro chi continua ad abusare dell'ambiente, ad esempio sperimentando il nucleare: sarebbe legittimare tacitamente gli eccessi degli altri Paesi. A nome del mio partito, impegno il Governo ad adempiere alle misure prescritte e chiedo al signor Presidente di ritenermi firmatario della mozione n.

tre rapporti ed un vertice che ancor di più hanno aggiunto forti elementi di preoccupazione per quanto riguarda la situazione del nostro pianeta. Vorrei ricordare innanzitutto l'allarme

aumentare. Sul banco degli imputati, e in questo il Rapporto ONU fotografa anche la situazione italiana, siede il settore dei trasporti responsabile di un aumento delle emissioni

ci presentano scenari assolutamente drammatici. Nel Rapporto si parla, inoltre, di 200 milioni di profughi a causa della distruzione di intere zone per siccità e alluvioni: una migrazione biblica che mai si era verificata nella storia. il Rapporto afferma anche con chiarezza che ormai non è più assolutamente prorogabile la necessità di individuare, con un nuovo Trattato, entro il prossimo anno, gli obiettivi più stringenti e uno sforzo internazionale per arrivare davvero a porre in atto atto politiche più incisive e più efficaci per cominciare a invertire la tendenza. Il terzo elemento è rappresentato dal Rapporto della FAO sullo stato di

non vi sono solo l'iniqua distribuzione delle risorse e le guerre, ma anche le catastrofi naturali (desertificazione, alluvioni) determinate dai cambiamenti climatici.

per il nostro Paese e non un fattore di perdita di occupazione, così come afferma la mozione presentata dal senatore Novi. apre una nuova finestra") *(UDC)*. Signor Presidente, nella mozione che abbiamo sottoscritto, sicuramente ispirata dalle migliori intenzioni, troviamo tante dichiarazioni di principio condivisibili. Tutti, nessuno escluso, escluso, abbiamo la giusta aspirazione a vivere in un mondo migliore, dove l'ambiente sia di qualità eccellente, dove i nostri figli possano crescere sani e forti. Il problema è che nessuno è disponibile a rinunciare al benessere acquisito grazie allo sviluppo industriale, uno sviluppo che spesso ha proceduto senza nessuna considerazione per l'ambiente e che rischia di danneggiare la qualità della nostra vita, senza dimenticare l'immensa mancanza di educazione che da sola ci imporrebbe il rispetto degli altri e dell'ambiente. Non è un problema solo momentaneo, come vediamo dalla gestione dei rifiuti in Campania, ma di tutto il Paese. Allora, credo io, dobbiamo essere realisti: molte volte la politica manca di questo. Dobbiamo darci degli obiettivi, ma questi obiettivi devono essere raggiungibili, altrimenti si cade nell'utopia. Solo una politica ambientale comune, oserei dire planetaria, può permettere il raggiungimento dello scopo; se così non fosse, l'unico risultato sarebbe quello di bloccare lo sviluppo del Paese, senza ottenere nessun beneficio dell'ambiente in senso generale. Importante, dunque, sarà il modo di procedere. Condividiamo che si chieda l'attuazione di politiche più incisive, che siano concordate in ambito internazionale, così come è necessario - e qui il Governo dovrà dare il meglio di sé - che si trovino gli strumenti per impegnare i Paesi più inquinanti ad essere sicuramente più virtuosi. Non dimentichiamo il fatto che i Paesi emergenti, proprio perché poco attenti al problema ambientale, oltre a quello della tutela dei lavoratori, si possono permettere di essere particolarmente aggressivi, operando in un contesto di concorrenza sleale verso gli altri produttori. Dunque, sì all'attuazione del Protocollo di Kyoto, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili. Così come condividiamo la necessità di intervenire, dando il via alla creazione di un circolo virtuoso che permetta alle famiglie un reale risparmio nel campo dell'energia, con il conseguente beneficio economico per le stesse. Siamo d'accordo sulla necessità di rafforzare la ricerca e fare del risparmio energetico una delle priorità, permettendo il rilancio della competitività del Paese e -consentitemi un po' di polemica - bisogna investire su questo, la finanziaria è anche il momento per farlo e mi sembra che questo Governo non sia stato particolarmente aggressivo. Così come crediamo veramente indispensabile il rapporto con l'impresa, principalmente con la media e la piccola, quella che costituisce la spina dorsale del nostro sistema produttivo ma che, proprio per il particolare dimensionamento, trova maggiori difficoltà ad investire in innovazione, rischiando di trovarsi fuori dal mercato. Dunque, non possiamo che condividere la mozione in esame. Ovviamente dall'azione che verrà intrapresa e da come sarà applicata nel nostro Paese, deriverà la nostra capacità chi poter essere protagonisti. Non dimentichiamo la situazione particolare in cui versa l'Italia nel campo energetico, ritrovandosi con un *gap*, rispetto agli altri Paesi, dovuto alla totale assenza dal settore nucleare. Una situazione che deve tenere conto del fatto che nel nostro portafoglio energetico la parte preponderante è svolta dal gas naturale, idroelettrico e olio combustibile. Proprio per questi motivi dobbiamo spingere, come giustamente riportato, per l'innovazione nel settore dei trasporti, della mobilità e della logistica. Dunque, nell'annunciare, come farò dopo, il voto favorevole dell'UDC, voglio ribadire la necessità di procedere *cum grano salis*. Lavoriamo per convincere tutti, ne siamo convinti, ma stiamo ben attenti a non procedere in modo solitario, facendone pagare al nostro mondo produttivo i costi senza ottenerne i necessari benefici perché, come bene sappiamo da Chernobyl in poi, non ci sono confini che possano fermare l'inquinamento. Non vorremmo azzerare il nostro, uscire dal processo produttivo e poi respirare l'aria inquinata prodotta da altri.

signori rappresentanti del Governo, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, ricordo bene la riunione di Rio de Janeiro, nella prima metà di giugno del 1992, quando ebbe luogo la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo L'immensa metropoli riceveva delegazioni governative di 175 Paesi, il maggiore evento internazionale fino ad allora conosciuto. Ma insieme a quelle arrivavano migliaia di persone da ogni parte del Pianeta in rappresentanza dei grandi sindacati dei lavoratori o di piccoli gruppi di produttori, Nazioni indigene con il loro sapere millenario, giovani studenti e vecchi scienziati. Aleggiava un arcobaleno sociale e si viveva in allegria e speranza. Da lì nasceva uno degli affluenti che pochi anni dopo avrebbe formato il generoso fiume del *Forum* sociale mondiale, più noto in Italia come il «movimento dei movimenti». Da quella riunione sbocciò il documento «Agenda 21», nel quale si promettevano la pace, lo sviluppo equilibrato e il rispetto della piccola casa comune: il pianeta Terra. I sogni si infransero contro il duro scoglio della globalizzazione neoliberale. Un modello di vita consumistico e illogico continuò crescere con ancora maggiore forza. La guerra tecnologica si perfezionò, con flotte di navi, sottomarini, aerei, carri armati, bombe sofisticate. Tutto ciò non solo spezza la vita di pochi combattenti considerati nemici e di molti civili innocenti, ma inquina la terra, i fiumi, i mari e lo spazio, consumando enormi quantità di energia. La destrutturazione di fabbriche, delocalizzate in vari punti del Globo, sempre in cerca di mano d'opera e materie prime più a buon mercato, fa sì che componenti di un prodotto viaggino migliaia di chilometri fino a che il prodotto stesso giunga alla sua fase finale e al punto di vendita. La controriforma agraria planetaria trasferisce i terreni fertili all'*agrobusiness* e distrugge la piccola agricoltura famigliare. Le foreste e i boschi sono divorati per fare spazio alle derrate del mercato mondiale, come la soia. Nei nostri supermercati si possono trovare manghi della Thailandia, avocado del Sudafrica, mele del Brasile o noci del Cile. Sono tutti prodotti ottimi, non ne dubito. Ma Ma una volta di più mi chiedo qual è il costo energetico di tutti questi trasporti (per tacere dei fertilizzanti, pesticidi o altro), mentre lo sforzo dovrebbe essere concentrato per la costruzione di un mercato interno nei Paesi più poveri e in generale per la realizzazione di una agricoltura destinata al consumo regionale, equilibrata, con bassi consumi energetici e chimici e con necessità contenuta di acqua. E questo vale anche per l'Italia. La ricerca di fonti alternative cammina con lentezza: gli scienziati, gli ecologisti, i movimenti sociali che denunciano le strade sbagliate imboccate dallo sviluppo neoliberale sono tacciati di essere visionari, arretrati, non riformisti, apocalittici. Ai giganteschi conglomerati scientifico-industriali non interessa un cambiamento di rotta, perché il dominio della riproduzione delle sementi, delle fonti di acqua, della ricerca militare, dei saperi in generale è una fonte enorme di profitto. Anche grandi scrittori di *bestseller* come Michael Crichton si adeguano alla linea di minimizzare i rischi, come dimostra il suo ultimo libro "Stato di paura". Ma nonostante tutto la realtà si sta imponendo. I pericoli che ci minacciano diventano patrimonio di milioni di esseri umani. Anche lo stesso presidente della Commissione dell'Unione Europea, José Manuel Barroso, nel confessare che probabilmente i Paesi dell'Unione Europea non rispetteranno la meta di riduzione di CO2, ha dichiarato: «Questo non è una elucubrazione di alcuni ecologisti, questo è un serio problema che minaccia il futuro della vita in questo Pianeta.» La riunione di Nairobi è importante e potrà fare rifiorire le speranze e segnare la storia umana e di tutta l'umanità. In questo senso voglio fare un appello direttamente al presidente Franco Marini, anche se non è presente in Aula in questo momento. Il Senato italiano non sarà rappresentato in questo incontro. Considero ciò una grave mancanza, come seria e dannosa per il Paese tutto è la costante non presenza di senatori italiani in altre riunioni internazionali. Si capisce il momento politico che viviamo con la esiguità della differenza di voti che separa i due blocchi. Chiedo, tuttavia, un intervento della Presidenza, affinché, usando la sua autorità e la sua capacità di mediazione, renda possibile l'auspicabile obiettivo che si riesca a compiere le missioni che fanno parte del nostro obbligo come senatori, a favore del prestigio dell'Italia. *(Applausi dai

il cambiamento climatico è una delle sfide più importanti che abbiamo davanti e pone gravi minacce alla prosperità e alla stabilità della nostra società. Il Protocollo di Kyoto tenta di fornire gli strumenti per raccogliere e vincere tale sfida, anche se la maggior parte dei Paesi industrializzati che sono vincolati ai suoi obiettivi sono in affanno. Sono in affanno perché i sistemi industriali mostrano vischiosità nel rispondere agli obiettivi posti; sono in affanno perché sullo sfondo vi è il grande problema energetico; sono in affanno nel riuscire a coniugare il binomio sviluppo e ambiente.

su quanto è stato fatto fino ad ora e a tessere la tela

per gli impegni che si dovranno prendere dopo il 2012. Oltre tale data scade, infatti, il Protocollo di Kyoto e le quote di emissioni dei Paesi coinvolti verranno rinegoziate. A Nairobi, però, non si arriva nel clima migliore. Il primo ministro canadese Harper ha definito, infatti, irragiungibili gli obiettivi e le scadenze dell'Accordo di Kyoto ed ha proposto un piano alternativo *made* *in* *Canada*. Dopo gli Stati Uniti, da soli responsabili del 36,1 per cento delle emissioni globali, e dopo l'Australia, vi è quindi il rischio di un'altra defezione importante che renderebbe sempre più complessa una concreta protezione del clima. Gli Stati Uniti d'America non hanno mai chiaro "no" a Kyoto, ma sostengono che il Protocollo è uno strumento della Convenzione sui cambiamenti climatici e, poiché loro ne fanno parte, non c'era bisogno, secondo il loro parere, del Protocollo di Kyoto. L'Europa è stata, e continua ad essere, un'apripista sul fronte dei cambiamenti climatici, ma da sola è responsabile solo del 14 delle emissioni globali di gas serra, e questa percentuale è destinata a diminuire con l'entrata sui mercati globali di Paesi come la Cina, l'India e il Brasile. Secondo il rapporto del 2005 sull'energia internazionale, se lo sviluppo di Cina, Brasile e India continuerà a questo ritmo in questi anni, nel 2030 avremo bisogno del 50 per cento in più di energia, determinando un aumento delle emissioni globali di CO2 pari al 55 per Di fronte a questo scenario, in cui l'Europa diventerà sempre più marginale sul palcoscenico globale delle emissioni, i Paesi dell'Unione Europea potranno avere invece un ruolo di primo piano, intensificando il lavoro diplomatico di pressione e persuasione nei confronti di quei Paesi che oggi non fanno parte della platea del Protocollo di Kyoto, ma che, dopo il 2012,

può decidere di andare avanti, ma deve essere consapevole che la sua battaglia solitaria avrà un impatto minimale sul fronte del cambiamenti climatici. Di qui al 2012, l'Europa al suo interno dovrà però svolgere la sua parte; dovrà considerare prioritariamente la convergenza delle politiche ambientali con quelle energetiche ed impegnarsi a sostenere finanziamenti ed incentivi a favore dell'efficienza energetica e delle fonti Proprio per avviare questa politica virtuosa, lo scorso anno alla Conferenza dell'ONU di Montreal sul clima è stato proposto dall'Italia di scorporare gli investimenti per Kyoto dal Patto di stabilità, un'iniziativa che ritengo debba essere

Il 19 dicembre del 2002 è stato approvato dal CIPE il Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra, aggiornato nel febbraio 2004, che prevede misure nazionali e di cooperazione tecnologica internazionale per centrare l'obiettivo di Kyoto. La legge finanziaria dello scorso anno ha previsto un primo stanziamento per Kyoto, rivolto soprattutto all'innovazione tecnologica: la diffusione della microgenerazione diffusa, le cosiddette centrali "fai da te", che a regime sarebbero in grado di ridurre le emissioni di CO2di 10 milioni di tonnellate all'anno, e l'idrogeno. La ricetta per centrare gli obiettivi di Kyoto è chiara a tutti e passa attraverso una minore dipendenza dai combustibili fossili, trasporti più puliti, efficienza e risparmio energetico e fonti alternative. Essa può rappresentare una grande occasione per rendere concreta la visione dell'ambiente come occasione di sviluppo. Le industrie, se sapranno cogliere quest'occasione, potranno diventare competitive sui mercati globali, ma non dobbiamo nasconderci che nel breve periodo l'applicazione del Protocollo costerà economicamente e si farà sentire anche sulle bollette elettriche.

il sistema europeo dell'*emission* *trading* in modo da evitare che settori industriali italiani ad alta efficienza paghino, attraverso l'acquisto di quote, lo sviluppo di settori europei meno efficienti. È necessario anche proseguire sulla strada dell'utilizzo dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo. I progetti di cooperazione internazionale, avviati soprattutto nei settori energetici, forestali ed industriali, consentiranno, ad esempio, di ottenere una riduzione di 60 milioni di tonnellate di anidride carbonica. La salvaguardia dell'ambiente - quindi, per quanto ci riguarda, le emissioni in atmosfera - non ha un colore politico e la firma della mozione n. 39, che è stata presentata qui, ne è la dimostrazione palmare. Non possiamo pensare di salvaguardare l'ambiente senza tener conto che dobbiamo anche far continuare ad esistere le nostre imprese che creano ricchezza e quindi occupazione. Su questi argomenti credo che non ci dobbiamo assolutamente dividere. Sviluppo sostenibile, termine coniato dalla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, vuole dire salvaguardia dell'ambiente, ma anche possibilità di far produrre ancora le nostre aziende. I cambiamenti culturali occorrono. L'ambiente non è solo un vincolo, come qualcuno sostiene (sempre meno per la verità); l'ambiente è anche un'opportunità. Quest'opportunità la dobbiamo cogliere anche attraverso la Conferenza internazionale dell'ONU, anche attraverso i cambiamenti climatici, anche attraverso una collaborazione più diretta di ordine internazionale. Se decidessimo, come Italia, ma anche come Europa, di adottare dei provvedimenti virtuosi che consentissero di non inquinare assolutamente, non avremmo comunque risolto il problema perché il problema non è nazionale e non è nemmeno europeo, ma è di carattere internazionale e mondiale. Insieme dobbiamo trovare il modo di raggiungere gli obiettivi. C'è un fatto però che mi fa essere ottimista: è cresciuta nel Paese e nel mondo la coscienza ambientale; è cresciuta in tutti, anche nel mondo imprenditoriale. Cogliamo l'occasione dell'accresciuta coscienza ambientale per mobilitarci anche dal punto di vista di un cambiamento culturale verso la salvaguardia dell'ambiente.

Ministro, la mozione n. 39 che stiamo discutendo è di fondamentale importanza innanzitutto per il merito, ma anche per il fatto che è stata sottoscritta dai senatori di entrambi gli schieramenti e ciò è raro in questo periodo

ne iniziano infatti ad osservare le conseguenze anche alle nostre latitudini. I fenomeni estremi diventano sempre più frequenti: dalle alluvioni che colpiscono l'Europa all'aumento impressionante del numero e della forza dei cicloni (il più famoso e devastante dei quali l'uragano Katrina, che colpì New Orleans un anno fa) che si formano nell'emisfero settentrionale del nostro pianeta. Complessivamente, come ricordiamo nella nostra mozione, i dieci anni più caldi mai registrati si sono avuti dal 1991 ad oggi. Ciò che ci deve più far riflettere, però, è una questione che assume anche una rilevanza etica. Le conseguenze più gravi dei cambiamenti climatici in atto le pagano infatti quei popoli, quelle persone, quegli uomini e quelle donne in carne ed ossa che non hanno alcuna responsabilità nell'aumento delle emissioni di gas serra che sono alla base, a loro volta, dell'incremento dell'effetto serra. Penso a quei milioni di profughi ambientali, spinti a scappare dalle proprie terre, divorate dalla desertificazione nell'Africa subsahariana. Ormai la comunità scientifica internazionale è praticamente unanime, a parte alcuni giapponesi spinti dalle *lobby* e non dalla scienza, nel dire che non sono le mucche sono le mucche di qualche Paese, ma le cause antropiche, il modo in cui produciamo e distribuiamo energia a causare l'aumento dell'effetto serra. Non era così appena dieci anni fa, quando vi era una battaglia anche nel mondo scientifico per affermare questa relazione causa-effetto, ma oggi questa è provata. Quindi, non possiamo più perdere tempo e dobbiamo imboccare con decisione la strada con la quale cambieremo il modo di produrre e distribuire energia, il modo in cui ci spostiamo, in cui si muovono le persone e le merci. Dobbiamo insomma responsabilmente, ed ovviamente con tutte le gradualità che non rendano velleitario questo percorso, incamminarci verso l'uscita dall'era del fossile. Yamani, lo storico ministro degli esteri dell'OPEC, usava dire che l'età della pietra non si concluse per l'esaurimento delle pietre, ma a causa dell'innovazione tecnologica. E così sarà per il petrolio. Infatti, Yamani proprio nell'innovazione tecnologica individuava il nemico mortale dell'OPEC. Su questo dobbiamo lavorare: risparmio energetico, inteso come politiche che stimolino l'efficienza energetica. Su questo per fortuna iniziano a vedersi i primi provvedimenti; penso a quello sull'edilizia già nella finanziaria attualmente in discussione alla Camera. Dobbiamo colmare un *gap* clamoroso che riguarda il nostro Paese rispetto all'Europa. Non è possibile che in Germania vi siano dieci volte più pale eoliche di quelle installate in Italia; non è possibile dire che nella fredda e piccola Austria vi siano 30 volte i pannelli solari che sono stati installati in Italia. Su questa strada dobbiamo marciare e su questa strada dobbiamo convincere il sistema economico italiano che si può scommettere per salvare il pianeta e per dare una *chance* anche le nostre imprese nella competizione globale. Un esempio per tutti è la STMicroelectronics di Pistorio che su questo ha fondato la sua capacità. Auspico, che la mozione che impegna il Governo su questa strada sia anche accompagnata dalla decisione del Governo di approvare finalmente il Piano nazionale delle assegnazioni,

di discussione e di conflitto, che pure si è registrata a volte su questi temi. Come peraltro sosteneva il senatore Matteoli, la battaglia contro il rischio di un cambio climatico sempre più preoccupante non dovrebbe trovare differenze di schieramento, bensì una convergenza unitaria perché il tema da affrontare è di gravità estrema

Vi sono tante sedi per parlare delle responsabilità. Oggi abbiamo bisogno di dare un segnale di cambiamento ancora più forte, ancora più intenso. Molti sono gli impegni che abbiamo preso, ma purtroppo, spesso e volentieri, alle dichiarazioni, tutte a favore della centralità ambientale, non seguono scelte conseguenti. Dobbiamo passare dalla sensibilità ambientale alla priorità ambientale. contrario, non riusciremo a fare le scelte necessarie. La sensibilità è cresciuta nell'opinione pubblica, in molti cittadini e in molte realtà dell'impresa, dell'economia e dell'informazione, ma la consapevolezza di quanto sia rilevante oggi questo tema è ancora scarsa.

parlamentari intervenuti, si può lavorare per sostenere le famiglie, perché ridurre il costo e lo spreco energetico riduce anche il costo delle bollette.

il cambio climatico possano aderire al Protocollo di Kyoto o, comunque lo vogliamo chiamare, a un serio protocollo per il taglio delle emissioni dei gas serra. Sappiamo infatti che gli appelli che si stanno sottoscrivendo a livello planetario non parlano di una riduzione del 6, del 7 o del 10 per di riduzioni del 30 o del 50 per cento nei prossimi decenni. La sfida è allora così alta che dobbiamo auspicare che tale impegno sia realizzato prima di registrare problemi di mutamento climatico più gravi. Lo scioglimento dei ghiacciai procede molto più velocemente di quanto ci si aspettava. La vicenda della Groenlandia o di quanto accade nella calotta polare artica è evidente, ma anche l'Italia ha problemi di cambio climatico. Noi viviamo il cambio climatico, abbiamo problemi nei ghiacciai delle Alpi; abbiamo un problema complessivo a fronte del quale saremmo degli irresponsabili se non intervenissimo. È evidente che Kyoto costa, ma quanto costa il cambio climatico? Quanto costa ogni centimetro di innalzamento del livello delle acque, in un Paese come questo, con 8.000 chilometri di coste, un'economia turistica e un notevole sviluppo di vita lungo le coste? La coalizione mondiale delle città di mare

delle emissioni italiane a 200 milioni di tonnellate, più 6 milioni che andranno all'asta, in modo che il ricavato venga riutilizzato per il risparmio e gli adempimenti del Protocollo di Kyoto.

inquinanti dal punto di vista della C02 e dei gas serra. Spero che da questo punto di vista riusciremo a trovare delle soluzioni. Un'ultima considerazione, che è anche un annuncio. Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ha deciso

«impegna il Governo ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di realizzare quanto già predisposto e in parte attuato dal Governo Berlusconi» - soltanto per motivi di tempo, perché

dalla maggioranza. Vediamo se lo schieramento cui appartengo si dividerà su questa mozione che riproduce quanto detto dall'allora Ministro dell'ambiente in Commissione.

è stato ratificato dai Paesi industrializzati, ad eccezione degli Stati Uniti e dell'Australia, e da molti Paesi in via di sviluppo. Secondo il Protocollo, soltanto i Paesi industrializzati devono ridurre le emissioni di gas serra, ma il loro impegno non sarà sufficiente per stabilizzare le concentrazioni atmosferiche a un livello non pericoloso, come richiesto dall'articolo 2 della Convenzione stessa. Entro il 2015-2020 le emissioni dei Paesi in via di sviluppo saranno uguali a quelle dei Paesi industrializzati. In occasione dell'ultima Conferenza sul clima, a Montreal, sono state avviate diverse discussioni al fine di coinvolgere tutti i Paesi nella riduzione delle emissioni. Si tratta, in particolare, dei Paesi «soglia» e dei Paesi le cui emissioni rappresentano una percentuale importante delle emissioni globali; in particolare, gli Stati Uniti e l'Australia che non hanno ratificato il Protocollo di Kyoto. Siamo quindi qui, perché dal 6 al 17 novembre a Nairobi si terrà la II Conferenza che vedrà coinvolti 157 Paesi che hanno a suo tempo ratificato il Protocollo di Kyoto e consentire così il proseguimento della discussione e del confronto apertosi a Montreal, ove era stato avviato un dialogo sulla collaborazione a lungo termine tra i Paesi al fine di esaminare apposite strategie che consentano agli stessi di partecipare agli impegni di riduzione dei gas serra. In particolare, ai Paesi in via di sviluppo che presentano le emissioni più elevate, cercando di individuare in maniera precisa gli obiettivi e gli impegni che ogni Paese aderente deve prefiggersi di perseguire attraverso politiche interne.

a far sì che il Governo s'impegni in modo attivo con altri Paesi firmatari e in sede europea affinché gli enunciati del Protocollo di Kyoto risultino effettivamente operanti. Non possiamo, infatti, ignorare le pesanti ripercussioni economiche e ambientali a cui andiamo incontro poiché ad oggi noi stessi non risultiamo essere stati ottemperanti alle quote assegnateci. Inoltre, fondamentale per un Paese come il nostro, a continuo rischio energetico, è la ricerca di fonti alternative rinnovabili che ci conducono a ridurre la nostra dipendenza dai combustibili di natura fossile, i quali, oggi come oggi, costituiscono la fonte energetica più dannosa per il nostro clima; senza contare poi il costo che in termini di bolletta ogni anno si riversa su tutte le famiglie italiane. L'impegno richiesto al Governo, soprattutto a livello di politiche interne, è prioritario e si richiede incisività e un grandissimo sforzo, anche di natura economica, per incentivare la ricerca e l'innovazione in settori in cui sino ad oggi risultiamo troppo mancanti e non per il livello dei nostri ricercatori, tra i più apprezzati nel mondo. L'impegno sarà quindi gravoso, ma i costi sarebbero ancora maggiori ove non si facesse nulla; del resto, è esattamente ciò che diceva il ministro Pecoraro Scanio poco fa. Essenziale è la collaborazione tra tutte le Nazioni affinché lo scenario a tinte fosche che si prospetta per il futuro delle nuove generazioni rimanga relegato alla fervida fantasia di qualche pittore. L'Italia può e deve svolgere un ruolo centrale; le ripercussioni economiche che si produrrebbero ove si lasci il dibattito in ambito scientifico sono quasi inimmaginabili, ma ancora di più a risentirne sarebbe la nostra salute e tutto l'ecosistema, già oramai compromesso da decenni di incuria e speculazioni. Consapevoli,

anzi richiediamo uno sforzo ancora maggiore al Governo, commisurato a un Paese come il nostro, un Paese in cui già da anni sono evidenti i segni delle manomissioni del territorio operate dall'uomo, ove si lamentano ogni inverno ingenti danni e anche vittime causate da nubifragi e inondazioni, un Paese che ha avuto già, quindi, un piccolissimo assaggio di cosa potrebbe verificarsi su scala mondiale. È notizia di questi giorni come i nostri ghiacciai siano ancora in fase di arretramento a causa del surriscaldamento globale. Esistono oggi tecnologie e studi per consentire una inversione di marcia al nostro pianeta. Quello di cui si necessita ora è la volontà politica ad operare questa inversione; è per tale motivo che oggi chiediamo al Governo di farsi portatore di questa coscienza del problema, di rendersi attore e non semplice spettatore in sede internazionale, di operare affinché queste non rimangano - come spesso accade - semplici parole, enunciati d'intenti.

per il quale in questo momento è riunita la Conferenza a Nairobi. Segnalo, anche da parte del nostro Gruppo, quella che consideravamo un'esigenza di rappresentatività della nostra Assemblea,

agli intenti condivisi da parte di tutte le forze politiche per un loro effettivo e coerente approccio in termini di soluzione sia sufficiente a dare un segnale, anche in quel lavoro internazionale, dell'interesse e dell'impegno dell'Italia per questa materia. Signor Presidente, il Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani voterà a favore

confortante, perché da parte un po' di tutti vi è stata la dichiarazione della necessità di una svolta decisiva e decisa per contrastare i cambiamenti climatici, sia a livello di impegni internazionali a Nairobi sia a livello nazionale. Voglio ringraziare il ministro Pecorario Scanio anche e soprattutto per la proposta, che qui ci ha presentato, di una Conferenza nazionale sul clima per il 2007, per dare il via ad un piano di misure

per la necessità, qui richiamata, di una conferenza nazionale del nostro Paese sull'energia. Il cambiamento climatico - come abbiamo visto - si manifesta, ormai, con evidenti segnali e rappresenta anche nel nostro Paese - non solo nei casi dell'Africa che citavo nel dibattito generale - una minaccia concreta per l'ambiente e per l'economia nazionale, in un territorio come il nostro, anch'esso soggetto alla desertificazione, alla siccità periodica, al dissesto idrogeologico. Contiamoli, questi costi, una volta per tutte, soprattutto per l'agricoltura, già sottoposta, oggi, a danni crescenti e al rischio di delocalizzazione per alcune delle colture più tipiche dell'area mediterranea. Dobbiamo, quindi, fare in modo che l'applicazione del Protocollo di Kyoto e le nuove misure per contrastare gli effetti del cambiamento climatico possano divenire divenire un fattore straordinario di competitività per l'economia del Paese e di crescita dell'occupazione. Su questo dobbiamo

termoelettrica; nei settori civile e terziario. Noi dobbiamo assolutamente ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili e Kyoto è una grande occasione

sostenibile, con ricadute benefiche sul piano ambientale nelle nostre città. Nel campo energetico è necessario fare dell'efficienza e del risparmio energetico, come recita la mozione, una vera e concreta priorità, con ricadute positive sul sistema produttivo e con un forte risparmio per le famiglie. E' necessario, però, investire seriamente con adeguate risorse nelle fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia, di calore, di biocarburanti attraverso un sistema vero, serio, incentivante, ma solo per le fonti rinnovabili. Basta alla truffa del finanziamento e degli incentivi alle fonti assimilate

per affrontare il secondo periodo, quello dal 2008 al 2012, con politiche più efficaci ed incisive, indispensabili per contrastare l'aumento delle emissioni.

con un grande sforzo grazie al quale l'innovazione tecnologica, gli investimenti, il cambio di cultura possono davvero offrire una nuova *chance* al nostro pianeta. Vorrei ricordare quanto stiamo già pagando in termini di biodiversità, quante specie vegetali ed animali

La Conferenza sul clima proposta dal ministro Pecoraro Scanio può essere l'occasione per un grande piano nazionale che traghetti l'Italia sulla nuova frontiera dell'innovazione, della ricerca e del vero miglioramento della qualità della vita del nostro Paese.

un immobilismo di quel Paese su tale tema. Ad ogni modo, il problema è sempre il solito: nessuno accetta di viaggiare a velocità diverse; dunque, dato che la necessità di interventi importanti comporta l'impiego di notevoli risorse, il rischio è che chi potrebbe fare di più non se la sente di impegnarsi a sacrificare il proprio sistema produttivo. L'Italia deve essere determinata nell'impegno, portando avanti con determinazione una politica seria per l'ambiente; una politica coerente che si assuma tutte le responsabilità, dallo Stato centrale fino all'ultima amministrazione comunale. Ritengo che le grandi politiche si possano attivare convincendo tutti:

Muoviamoci subito, troppi sono i mezzi pesanti che inquinano spudoratamente senza l'intervento di nessuno: questo è solo un piccolo esempio. Oggi in tanti ci ritroviamo d'accordo su un impegno importante, non lasciamolo cadere, non lasciamo che passi l'idea che la colpa è sempre degli altri! L'ambiente è di tutti, specialmente di chi verrà dopo di noi! Con il voto favorevole sulla mozione a prima firma del senatore Ronchi, l'UDC si assume la propria responsabilità e prende un impegno formale, speriamo si possa continuare tutti insieme.

e l'indirizzo politico nei confronti della Conferenza delle parti di Nairobi. Faccio questo con grande convinzione a nome del Gruppo al quale appartengo; con la stessa persuasione oggi esortiamo il Governo a colmare il grave divario nell'attuazione degli impegni del Protocollo di Kyoto. Seppur limitato nei suoi scopi, tale accordo ha rappresentato e rappresenta tuttora una fondamentale pietra angolare nella *governance* ambientale globale multilaterale, sempre in bilico tra unilateralismo e approccio esclusivamente volontario. Il *mix* di politiche pubbliche, vincoli e approccio di mercato avrebbe dovuto garantire una gestione ottimale del bene comune aria. A Nairobi si farà un bilancio e si cercherà di discutere anche del dopo Kyoto, cioè cosa la comunità internazionale dovrà fare dal 2012 in poi per ovviare ai ritardi e alle lacune anche congenite all'approccio del Protocollo di Kyoto. Proprio per questo crediamo che sia oggi occasione di fare un bilancio, ma anche di cominciare a guardare avanti, cercando di elaborare strategie e approcci innovativi che diano un assetto più equo e partecipato alla necessità di mitigare l'emissione di gas serra e tutelare l'atmosfera globale. Riteniamo che ciò possa essere possibile soltanto attraverso il riconoscimento e la restituzione del debito ecologico che il Nord ricco del pianeta ha nei confronti dei Sud impoveriti e sottosviluppati. Dobbiamo fare un passo in avanti ed abbandonare le suggestioni relative all'introduzione di innovazioni tecnologiche come unica via d'uscita per rendere il nostro modello di sviluppo compatibile con gli imperativi ecologici. Non ci illudiamo: il modello economico fondato sulla crescita quantitativa non è conciliabile con la finitezza della biosfera, checché ne dica anche il rapporto Stern che continua a pensare che la crescita economica possa essere compatibile con la necessità di ridurre e stabilizzare l'emissione di gas serra. Riteniamo opportuno praticare un nuovo approccio che metta al centro la giustizia economica ed ecologica globale e riconosca che l'aria (come l'acqua, la terra e i saperi) sia da considerare come un bene comune. Un approccio equo, quindi, fissa il principio che l'atmosfera e l'aria non sono prodotti di mercato, ma beni comuni che forniscono beni pubblici globali e quindi andrà riconosciuto il principio del diritto di ognuno, ogni abitante della terra, ad una eguale quota di atmosfera. Ne consegue dunque che i Paesi industrializzati hanno già sovrautilizzato le loro quote di emissione, generando un debito di carbonio, un debito ecologico, superiore al debito economico che i Paesi indebitati e poveri hanno nei confronti dei nostri Paesi del G8 e via dicendo. Condividiamo quindi le preoccupazioni dei movimenti sociali e delle associazioni ambientaliste di tutto il mondo che oggi chiedono giustizia climatica ed affermano che il commercio di permessi di emissione non fa altro che rafforzare le diseguaglianze sociali in varia forma. Gli effetti dei mutamenti climatici rappresentano, infatti, una grave violazione dei diritti umani e anche sono fonte e possibile causa di future guerre, come sottolineato di recente in un importante studio dell'*Oxford* *Research Center* intitolato «Sicurezza sostenibile per il XXI secolo». I meccanismi di sviluppo pulito previsti dal Protocollo di Kyoto permettono poi che si continui a esplorare, sfruttare e bruciare le riserve fossili del pianeta. Altro effetto perverso è la privatizzazione di acqua e terra, fonti di sostentamento delle comunità locali e contadine, attraverso piantagioni industriali di alberi o grandi dighe. Il secondo tema riguarda il ruolo della Banca mondiale nel dopo Kyoto. Il comunicato finale del G8 di San Pietroburgo riafferma l'incarico già dato al G8 di Gleneagles a questa istituzione finanziaria, incaricata appunto di creare un nuovo quadro di riferimento per le energie pulite e lo sviluppo, incluse le questioni di investimenti e finanziamenti. Un'incongruenza: la Banca mondiale, infatti, prevede di continuare ad investire almeno 10 miliardi di dollari nei prossimi anni in combustibili fossili, contraddicendo quindi questo mandato politico e perpetuando un bilancio negativo nella gestione delle risorse naturali e nella riduzione delle emissioni di gas serra associate ai suoi progetti. Chiediamo pertanto che l'Italia a Nairobi, e anche oltre, metta in discussione il ruolo centrale della Banca mondiale. In conclusione, pensiamo che il Governo italiano possa fare molto, dovrà fare molto, continuerà a fare molto e certamente dovrà impegnarsi ancor di più a soddisfare gli impegni presi a Kyoto ma anche a sostenere, a nostro parere, una necessaria inversione di rotta anche nella filosofia di fondo, nella cultura che riguarda le questioni ambientali globali, per coniugare finalmente sostenibilità, equità e giustizia sociale ed economica. Grazie, Presidente, Alleanza Nazionale voterà la mozione a firma dei senatori Ronchi, Matteoli ed altri, nella convinzione che la via tracciata dal Protocollo di Kyoto rappresenti una strada obbligata per affrontare la sfida che il cambiamento climatico in atto ha lanciato all'intera comunità internazionale. Alleanza Nazionale esprimerà questo voto nel solco di quel percorso virtuoso che ha visto l'Italia negli anni 2001-2006 fattivamente operare per dare concreta attuazione agli accordi protocollari, attraverso interventi rilevanti sia sul piano nazionale che internazionale, con particolare attenzione rivolta all'innovazione e alla cooperazione tecnologica. Lo farà, peraltro, ben sapendo che la sfida climatica, per avere possibilità di vittoria, deve essere affrontata al di là di ogni deriva ideologica, con assoluto realismo e nella consapevolezza che sia indispensabile per l'Italia e l'Europa non solo e non tanto operare al proprio interno per ottemperare integralmente alle previsioni protocollari ma anche e soprattutto adottare ogni opportuna iniziativa, diplomatica e politica, per coinvolgere concretamente quei colossi dell'economia, sia tradizionali, quali gli Stati Uniti d'America, sia emergenti, come Cina, India e Brasile, che da soli sono responsabili della quasi totalità delle emissioni inquinanti. Senza questo concreto coinvolgimento, infatti, gli sforzi italiani ed europei saranno pressoché completamente vanificati, con una ulteriore ed ingiustificata penalizzazione non solo in sede internazionale ma anche continentale del nostro sistema imprenditoriale, che già gode, anche rispetto agli altri Paesi europei, di una più alta efficienza energetica e che quindi, senza alcun positivo ritorno sul piano ambientale, patirebbe una insostenibile perdita di competitività. Oggi non serve, dunque, raschiare ancora il fondo del barile in Italia, con una criticabile mentalità da primi della classe, ma soprattutto dare effettivo impulso a tutti quei meccanismi flessibili che, attraverso i progetti di cooperazione, permettono di ridurre le emissioni in altri Paesi, infinitamente più inquinanti del nostro. Con tale consapevolezza e nella profonda convinzione che questa - e non altre - sia l'unica strada percorribile, Alleanza Nazionale voterà a favore

risolverle con un grande spirito di realismo e di umiltà, senza ricorrere o rifarsi a culture tipiche del fondamentalismo ambientalista. Sappiamo - e sono dati certi - che le letture dei satelliti negli strati più bassi della troposfera non indicano alcun aumento della temperatura da ventitré anni a questa parte. Sto parlando delle letture dei satelliti. I dati climatici della Terra negli ultimi 1.000 anni dicono anche che il XX non è stato il secolo più caldo. 5.000 anni fa - a proposito di effetto serra e di riscaldamento - in Italia vivevano elefanti, gazzelle, antilopi. Il *record* degli anni più caldi Il *record* degli anni più caldi spetterebbe ai cinque secoli medievali, compresi tra l'800 e il 1300. Nel Medioevo in Inghilterra si coltivava la vite e la Groenlandia era libera da ghiacci.

Ora il fondamentalismo verde vorrebbe negare queste realtà scientifiche e accertate. Ciò non significa che il Protocollo di Kyoto non debba trovare applicazione. Significa, però, che bisogna prendere atto che il Protocollo di Kyoto non basta. Grandi Paesi in via d'industrializzazione, come la Cina e l'India, che da soli già oggi emettono il 30 per cento di gas inquinanti ad effetto serra, non hanno sottoscritto il Protocollo di Kyoto. Un Paese come il Brasile, il Brasile, che ospitò la famosa Conferenza di Rio, nella quale fu lanciato il tema dello sviluppo sostenibile, non ha ancora aderito. Non hanno ancora aderito altri Paesi, come gli Stati Uniti. La Russia ha aderito soltanto perché può vendere sul mercato delle emissioni i suoi crediti. La Russia,

da Paesi terzi, come il Marocco o la Russia, il diritto ad inquinare, cioè il diritto ad emettere i gas serra. Con l'intervento di quei Paesi si compensa il gas serra emesso dal nostro Paese. Signor Presidente,

interno: con le politiche del Ministero dell'ambiente, tale Governo ha fatto sì che il Protocollo trovasse attuazione con impegni concreti, coinvolgendo anche le imprese e la società civile portando avanti anche una politica di nuova pedagogia ambientalista. La mia mozione, in realtà, voleva rivendicare la specificità delle politiche ambientali del Governo Berlusconi, ma, siccome non intendo provocare divaricazioni nelle posizioni all'interno dei Gruppi del centro‑destra, la ritiro. Nessuno mi Nessuno mi può impedire, però, di esprimere il mio dissenso verso la mozione che quest'Aula approverà quasi all'unanimità.

Il perché a me sembra abbastanza chiaro. Con la globalizzazione si immettono nel mercato globale miliardi di nuove persone. Le economie di questi Paesi, come quelle dei Paesi industrializzati, si basano, per la gran parte, sull'uso di combustibili fossili, che si chiamano così proprio perché generati nell'era fossile. In poche centinaia di anni, e con un'accelerazione in questo decennio, stiamo liberando miliardi di tonnellate di anidride carbonica contenuta nei combustibili fossili, provocando uno sconvolgimento globale del clima.

infatti, qualora fosse interamente realizzato, comporterebbe una riduzione solo del 5,2 per cento rispetto alle emissioni del 1990, non è sufficiente. Un conto però è dire che esso non è sufficiente per tornare indietro; altro è sostenere che non è sufficiente per fare un passo ulteriore. È verissimo - lo sottolineava anche il collega Matteoli dobbiamo puntare a un coinvolgimento più forte degli Stati Uniti d'America. Anch'io sono ottimista perché alcuni Stati, all'interno degli Stati Uniti, hanno già sottoscritto impegni anche più stringenti di quelli previsti dal Protocollo di Kyoto come impegno statale,

i Paesi in via di sviluppo, i cosiddetti Paesi non-annesso, che non hanno ancora assunto impegni quantificati di riduzione delle emissioni: questo è il punto.

Per quanto riguarda l'Italia, bisogna utilizzare anche qui l'occasione del Protocollo di Kyoto per l'innovazione del sistema produttivo produttivo e del sistema energetico come occasione di nuova qualità dello sviluppo. Ma chi, più dell'Italia, ha interesse a ridurre l'uso dei combustibili fossili? Noi siamo grandi importatori di combustibili fossili e questo costa all'economia nazionale una bolletta energetica che, ad esempio, nel 2005 euro. C'è una convergenza economico-ambientale nelle politiche del Protocollo di Kyoto: usare meno fossili, promuovere efficienza, usi appropriati, risparmio e tutte le fonti rinnovabili possibili. Mi pare che su questa ricetta si registri un'ampia convergenza in quest'Assemblea. richiederà delle traduzioni operative - ritengo - anche più efficaci. Alcune sono state annunciate ed alcune sono anche previste nella finanziaria. Credo però che in questa direzione bisogna accelerare. Apprezzo anch'io l'annuncio fatto dal ministro Pecoraro Scanio di una Conferenza nazionale sul clima. Spero che ciò diventi un'occasione di coordinamento delle politiche. Adesso si avverte la necessità di integrazione forte fra le politiche energetiche e ambientali, fra le politiche dei trasporti e le politiche dell'efficienza energetica, fra le politiche della generazione distribuita, fra le politiche agro-energetiche. Si tratta di occasioni di sviluppo e di occupazione, altro che Protocollo di Kyoto che provoca 250.000 disoccupati! Il Protocollo di Kyoto può essere subìto come un costo, ma può anche essere occasione di investimento e di innovazione. Il Governo inglese ha affidato a una Commissione, presieduta da *sir* Stern, un rapporto di studio internazionale sui costi e le opportunità contenute negli investimenti delle politiche e delle misure per il cambiamento climatico su scala globale. È interessante vedere da questo primo rapporto globale in tal senso (rapporto Stern) come, da una parte, mancate politiche hanno dei costi; mancate politiche e misure hanno dei costi anche economici, oltre che sociali e ambientali in relazione al cambiamento climatico; mentre, dall'altra, l'attuazione su scala globale delle politiche e delle misure del Protocollo di Kyoto può addirittura accelerare la qualità e la crescita su scala globale, offrendo nuove opportunità di investimento, di innovazione tecnologica, nuovi tipi di produzione e di consumo. Insomma, una sfida che abbiamo di fronte. Credo che la convergenza ampia realizzata al Senato renda l'Italia più forte sulla scena internazionale su questo tema; ci dia anche più forza su politiche e misure per affrontare questa grave crisi climatica globale e rappresenti anche una nuova opportunità per l'Italia e penso anche per l'Europa.

contemporaneamente dell'XI Conferenza delle parti che hanno ratificato la Convenzione sui cambiamenti climatici costituiscono due occasioni importanti per cercare di dare un'accelerazione a quel processo multiforme che aggancia parecchi settori della nostra convivenza sociale, affinché l'obiettivo della riduzione dell'8 dell'inquinamento fissato dal Protocollo di Kyoto possa essere raggiunto o comunque approssimato il più possibile. Sappiamo che non tutti i Paesi del nostro del nostro globo sono su questa posizione. Sappiamo che gli Stati Uniti e i Paesi in via di sviluppo, hanno reticenze, per tutelare il loro sviluppo economico, ad osservare norme di comportamento che possono dare

Noi riteniamo, però, che vi sia la possibilità anche di un impegno interno del nostro Paese per accelerare il più possibile per andare incontro a questi obiettivi che saranno affrontati nelle due Conferenze. Diceva il collega Libè del problema dei trasporti; altri parlavano del problema del risparmio energetico che deve diventare un'effettiva priorità. Sottolineiamo tutto questo e lo condividiamo. Ecco perché, Presidente,

ha approvato il mantenimento in servizio sino al 31 ottobre 2006 di 1.316 agenti ausiliari di leva del 63° e 64° corso allievi che ne avessero fatto domanda. su sollecitazione dello stesso Parlamento, assunse l'impegno a ulteriormente prorogare tale permanenza in servizio per non generare pericolosi vuoti nell'apparato della pubblica sicurezza, che peraltro non potrebbero essere altrimenti riempiti in un momento di grande impegno dello Stato nel contrasto al terrorismo ed al crimine organizzato. La spesa prevista dal comma 2, nella misura di 8.650.000 euro, fa riferimento ai soli salari, trattandosi di personale già pienamente impiegato in attività di servizio. Unica novità è l'introduzione alla Camera dell'articolo 1-*bis*, che autorizza il trattenimento in servizio a domanda, sino al 31 dicembre 2006, degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico che abbiano terminato senza demerito l'ulteriore ferma annuale. Signor Presidente, anche in questo caso è stata prevista una spesa con un vincolo di bilancio a non oltrepassarla. Non vi è stato alcuna dibattito durante l'*iter* in Commissione, poiché ha registrato la piena approvazione di tutta la Commissione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo dinanzi alla conversione in legge di un decreto teso a prorogare fino a fine anno la presenza di 1.316 allievi ausiliari della Polizia di Stato. Si tratta degli ultimi agenti provenienti dal soppresso servizio di leva e senza tale intervento questi giovani, dopo oltre due anni di formazione ed esperienza, sarebbero stati congedati a ottobre. Esprimo un giudizio favorevole sul provvedimento perché ritengo urgente affrontare tutte le situazioni di precariato nella pubblica amministrazione. La stessa grande e bellissima manifestazione di sabato contro la precarietà ha evidenziato come questo grave fenomeno riguardi una grande massa di giovani, ma non solo giovani, impossibilitati a costruirsi un futuro e costretti a continuare a vivere nell'insicurezza, non solo economica. In particolare, la precarietà nell'amministrazione dello Stato - e segnatamente nelle forze dell'ordine - è un dato recentissimo che riprende una pratica, in vigore sino alla riforma della pubblica sicurezza del 1981, quale sistema di controllo generalizzato delle gerarchie sui lavoratori. Tale dato dovrebbe preoccupare tutte le forze politiche perché, oltre a determinare situazioni di incertezza, di frustrazione nel lavoratore, lo sottopone al controllo totale ed indiscriminato della gerarchia. Il problema del sott'organico delle forze dell'ordine non può trovare certamente risposta solo da questo decreto, ma in sede di esame della finanziaria si devono trovare le risorse in grado di dare stabilizzazione al lavoro degli operatori del settore: in particolare, va prevista l'immissione nei ruoli degli ausiliari anche di altri Corpi - penso, ad esempio, al servizio dei Vigili del fuoco, al Corpo forestale dello Stato, alla Polizia penitenziaria - in servizio da anni dopo i vari corsi di formazione. La legge finanziaria - in particolare all'articolo 57 - deve programmare dunque un numero adeguato di personale nelle forze di polizia per il triennio 2007-2009, prevedere lo stanziamento di risorse per il rinnovo contrattuale e il ripristino delle norme ingiustamente soppresse relative al rimborso delle spese sanitarie sostenute per infermità da causa di servizio. Più in generale, ritengo che il Governo dovrà prevedere la costituzione di un tavolo tecnico destinato a costruire un progetto complessivo...

La situazione della sicurezza in Italia è, infatti, paradossale: con un numero di addetti e un livello di spesa simili agli altri Paesi europei, si ottengono risultati insoddisfacenti, sia per i cittadini che per gli operatori del settore. Servono strumenti tecnologicamente avanzati per analizzare vecchie e nuove illegalità; servono investimenti adeguati a tale riguardo. Ma spesso i problemi più frequenti nel controllo del territorio riguardano l'organizzazione delle risorse umane e finanziarie, utilizzate in modo spesso irrazionale, con duplicazioni e sovrapposizioni. Manca il personale dove ve ne sarebbe più bisogno, i materiali essenziali sono insufficienti, gli strumenti tecnologici inadeguati. I tagli effettuati al settore dalle precedenti finanziarie hanno determinato situazioni di disagio. Cito solo due esempi, signor Presidente: a Palermo si è costretti a togliere le auto blindate a chi è impegnato in prima linea nella lotta alla mafia; a Roma sono state tagliate del 50 per cento le risorse umane e i mezzi del reparto volanti della Polizia. Il massimo impegno va concentrato in stretta cooperazione con le istituzioni locali e la società civile - nel contrasto alla criminalità organizzata, che nei nostri territori soffoca la vita civile, ostacola l'esercizio dei diritti infiltrandosi nelle istituzioni e nella vita economica. Si dice che tra i cittadini è diffusa la richiesta di maggiore sicurezza. Pur tralasciando di sottolineare come i mezzi di informazione hanno in questi anni giocato un ruolo determinante nell'amplificare le paure dei cittadini (rivolte ad esempio alla presenza dei migranti nel nostro Paese) c'è certamente bisogno di sicurezza nelle nostre strade, nei luoghi più vicini ai cittadini, ma anche in settori spesso trascurati che riguardano la sicurezza nei luoghi di lavoro, la repressione del lavoro nero, l'azione nei confronti dei danni ambientali, degli abusivismi, dell'evasione fiscale, dell'usura e - soprattutto - nei confronti della violenza contro i minori e le donne. Ma l'intervento repressivo non è efficace se non viene affiancato da un complesso adeguato di politiche sociali. Ritengo che il Governo dovrà opportunamente prevedere la costituzione di un fondo speciale presso il Ministero dell'interno per far fronte alle emergenze, quale ad esempio in questi giorni vediamo nella città di Napoli. In questa città stiamo assistendo, in queste ultime settimane, a una preoccupante *escalation* di crimini gravi concentrati nello spazio di pochi giorni. Anche se le statistiche annuali relative ai reati non evidenziano complessivamente un incremento del fenomeno, occorre senz'altro intraprendere misure adeguate da parte del Governo, con un impegno più mirato e organizzato rispetto al passato per far fronte a questa grave situazione. Il ministro Amato sta predisponendo un piano di interventi, ne discuteremo approfonditamente i dettagli nei prossimi giorni, ma non possiamo non evidenziare alcuni aspetti strutturali gravi che lo Stato deve affrontare con politiche adeguate, non certamente concentrate sugli aspetti relativi alla sicurezza. I tagli agli enti locali hanno comportato una grave carenza di politiche economiche e di sviluppo per il Mezzogiorno che ha incrementato le disuguaglianze territoriali. A Napoli i problemi veri riguardano il lavoro, la povertà, la scuola. Fino a pochi anni fa esistevano le grandi aziende (come l'Ansaldo, l'ILVA, l'Aeritalia), c'era una parte importante del tessuto sociale costituito da operai, dirigenti. Ora non più, non c'è speranza di lavoro stabile, nell'assenza quasi totale di una seria politica industriale. Si è diffusa la povertà, l'insicurezza. La camorra ha avuto, nel tempo, una funzione

Non serve l'esercito a Napoli, non serve schierare le truppe agli angoli delle strade. Non si deve sfruttare il desiderio di sicurezza dei cittadini per militarizzare il territorio. L'insicurezza si combatte ricostruendo il tessuto sociale. Quando si colpisce la criminalità si sta certamente liberando il territorio, ma se poi non lo si occupa con diritti, lavoro, servizi, cultura, lo rioccupa la camorra. Un terzo della popolazione napoletana è rappresentata da giovani: è la fascia più colpita dall'insicurezza sociale e dalla precarietà. Assistiamo ad una vera e propria disgregazione sociale: in questi giorni, per occupare un marciapiede o per una ragazza, dei minorenni hanno anche ucciso. La vita ha perso valore. Chi li spinge a impiegare bene le loro potenzialità, a esigere i propri diritti, oltre a compiere i loro doveri? A Napoli solo l'1 per cento delle scuole sono a tempo pieno, contro l'88 per cento di Milano. L'emergenza Napoli si combatte anche e soprattutto a scuola, perché ciò può sottrarre tempo alla strada, incrementa la formazione della persona e la sua educazione alla legalità. Negli istituti si assiste a un abbandono scolastico che sfiora il 50 per cento. Lo scorso anno oltre 10.000 ragazzi - per la maggior parte ragazzini delle scuole medie - hanno abbandonato gli studi. Non hanno alcun futuro: la maggior parte prende la strada del lavoro nero, una parte entra nel giro della microcriminalità. Soltanto ieri i telegiornali riferivano che i nuovi *boss* assoldano i ragazzini a 500 euro a settimana! Occorre dare risposte al disagio crescente battendo la disperazione che spesso si unisce all'ansia di trovare facilmente denaro. Dobbiamo far funzionare le istituzioni, le scuole, favorire l'associazionismo. Invece, di provvedere agli strumenti in grado di affrontare questi gravi aspetti strutturali, i problemi di bilancio hanno sempre più spinto verso i tagli delle risorse alla scuola, ai servizi degli enti locali, alla macchina della giustizia. A questo proposito, solo ieri è stato lanciato l'allarme da parte dei magistrati: per riportare la legalità, oltre alla sicurezza va garantita la velocità della giustizia, occorre dare maggiori risorse e dignità del lavoro a questa istituzione. Concludo, signor Presidente e onorevoli colleghi, esprimendo il giudizio favorevole di Rifondazione Comunista al decreto-legge oggi in esame, nell'augurio che la situazione sociale che emerge dai nostri territori spinga spinga questo Governo a non limitarsi ad adottare provvedimenti tampone, come questo che limita i suoi effetti al 31 dicembre, ma ad affrontare la crisi con provvedimenti organici e soprattutto condivisi e partecipati

il tema dell'ordine e della sicurezza pubblica, mai come in questi ultimi tempi, balza agli occhi in maniera lampante: siamo di fronte ad una delle problematiche del nostro Paese più sentite dai cittadini. I nostri cittadini, in special modo quelli della città di Napoli, vivono quotidianamente una realtà in cui la micro e la macrocriminalità imperano, vivono nell'insicurezza e nella paura: lo Stato ha il dovere di non abbandonarli, di rassicurarli. Lo Stato ha il dovere di far sentire che c'è! La problematica dell'ordine e della sicurezza pubblica necessita, dunque, di essere affrontato dal Governo con un impegno assolutamente straordinario e con misure idonee. Oggi ci troviamo ad esprimere il nostro voto per garantire la conversione in legge di un decreto che va nella giusta direzione. Consente, infatti, di non sguarnire la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri di unità di personale importanti che oggi sono al servizio del Paese per contrastare la criminalità. È decisamente importante non far venire meno, proprio in un momento in cui lo Stato sta affrontando una tragica emergenza, la possibilità concreta per le forze dell'ordine di avere al proprio interno, nel proprio organico, un notevole numero di persone. Il decreto che ci accingiamo a votare costituisce però solo un piccolo, seppur concreto, passo di un percorso articolato di misure durature che il Governo dovrà sostenere per la lotta alla criminalità. Le norme in questione, infatti, prorogano fino al 31 dicembre 2006 la presenza di 1.316 agenti ausiliari della Polizia di Stato, appartenenti al 63° e 64° corso di allievo agente ausiliario di leva, e di circa 400 ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, frequentatori del 1° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri. Le suddette norme avranno, quindi, scadenza il 31 dicembre prossimo. È dunque assolutamente opportuno, affinché le misure urgenti del decreto-legge non risultino nei fatti assolutamente inefficaci, attirare l'attenzione del Governo sull'opportunità e sulla necessità di intervenire adeguatamente nella legge finanziaria per dare continuità alle norme in oggetto ben oltre la data indicata nel decreto. Spero vivamente, pertanto, che la Camera accolga la proposta emendativa del relatore di maggioranza al testo dell'articolo 57 del disegno di legge finanziaria (che attualmente prevede l'assunzione solo di 1.000 unità per le forze di polizia), volta ad autorizzare l'assunzione di 2.000 agenti di Polizia. Di questi, 1.326 sarebbero proprio gli agenti trattenuti in servizio dopo il periodo di leva oggetto del decreto al nostro esame. L'obiettivo della disposizione è proprio quello di evitare la creazione di precariato nelle forze di polizia, specie - lo voglio ribadire chiaramente - in un momento in cui occorre un forte e copioso dispiegamento delle forze di pubblica sicurezza in territori piagati dal male intestino della microcriminalità e della criminalità organizzata; criminalità che sta generando gravi conseguenze sociali e psicologiche, come la limitazione dei comportamenti e dei movimenti delle persone. I cittadini napoletani hanno il diritto di vivere una vita normale! Altro emendamento annunciato al testo della finanziaria che dovrà trovare necessariamente accoglimento, sempre al fine di poter garantire la piena e concreta funzionalità dell'amministrazione della pubblica sicurezza per consentire un adeguato controllo del territorio, è quello riguardante l'aumento di 29 milioni di euro alle dotazioni dei Carabinieri e di altri 29 milioni a quelle della Guardia di finanza.

poiché risponde, seppur non fornendo una misura di carattere strutturale che la maggioranza esprimerà - ne sono certo - in sede di legge finanziaria, all'intendimento per cui la sicurezza è un bene sociale che lo Stato deve riconoscere responsabilmente, fornendo risposte consapevoli ed efficaci a fronte di una crescente domanda che proviene dalle nostre comunità. *(Applausi

che risolve un problema sentito dai giovani allievi ufficiali dei carabinieri ausiliari del ruolo speciale, la cui professionalità acquisita nei corsi cui hanno partecipato è utile e resta al servizio della sicurezza del nostro Paese.

arruolati nel 1999, dopo aver svolto il servizio di leva, la ferma biennale ed un ulteriore periodo di richiamo che per taluni è durato fino a diciotto mesi. Dopo tale periodo non furono raffermati nonostante fossero stati dichiarati idonei dopo regolare concorso, perché su di loro ebbero la precedenza per l'accesso all'Arma dei carabinieri i volontari delle altre Forze armate. Dal 2006 ai volontari delle Forze armate sarà riservato il 100 per cento dei posti per arruolamento nell'Arma dei carabinieri e nelle altre forze di polizia; ciò comporta l'impossibilità per qualsiasi cittadino che non abbia prestato servizio come volontario in ferma prefissata nelle Forze armate di partecipare a concorsi per arruolamento nelle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Secondo la vigente normativa, inoltre, per partecipare ai concorsi per volontari occorre non aver superato il 25° anno di età; i succitati 300 carabinieri, 300 carabinieri, essendo stati arruolati nel 1999 e congedati nel 2003, dopo quattro anni, hanno quasi tutti superato tale limite di età. ad essi la preclusa la possibilità di tentare di rientrare nelle forze di polizia tramite i concorsi previsti per l'arruolamento dei volontari, cioè tramite la normativa intervenuta al loro congedo. L'ordine del giorno G2 si propone, quindi, di impegnare il Governo affinché predisponga «le opportune iniziative», che permettano «ai Carabinieri ausiliari congedati da non più di quattro anni di partecipare a concorsi che consentano la loro riammissione in servizio anche superando i vincoli relativi ai limiti di età». Stiamo avanzando,

alla loro prestazione in servizio definiti. È del tutto evidente, inoltre, che si tratta di una proposta che consente di operare considerevoli risparmi, anche sui costi di formazione e addestramento, trattandosi di Carabinieri dei quali è già stata accertata e sperimentata l'idoneità al servizio dell'Arma. Per quanto riguarda G3, va ricordato che nel 2004 sono stati indetti concorsi «per il reclutamento di 177 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni dell'esercito, di 24 Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo Commissariato ed Amministrazione dell'Esercito, di 24 Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti». Il Ministero della difesa, nell'ambito delle misure sul risparmio previste dalla legge finanziaria, ha ridotto in un secondo momento il numero dei posti messi a concorso: «la Direzione generale del personale militare del Ministero della difesa, con decreto dirigenziale del 31 dicembre 2004 e successivi provvedimenti, ha dichiarato idonei e vincitori dei suddetti concorsi solo 38 ufficiali, di cui 30 del concorso relativo a 177 sottotenenti delle Armi, 4 del concorso relativo ai 24 sottotenenti del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e 4 del concorso relativo ai 24 del Corpo di commissariato e amministrazione, negando ad altrettanti 38 ufficiali, idonei ed anch'essi vincitori dei concorsi in questione, il passaggio in servizio permanente; la succitata Direzione generale», successivamente, per coprire vacanze organiche, «ha indetto nel 2005 e nel 2006 nuovi concorsi per il reclutamento di Sottotenenti in servizio permanente, per i quali, a quanto risulta, l'elenco dei possibili vincitori non coprirebbe il numero dei posti messi a concorso». Questa è stata considerata una vera e propria ingiustizia da parte dei vincitori del concorso, che richiedevano di essere riassorbiti prima di bandire nuovi concorsi, anche perché la mancata assunzione derivava solo dal taglio delle risorse. Conclusivamente, signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo - che, lo vedo, ne segue con attenzione le motivazioni - l'ordine del giorno G3 si propone di impegnare il Governo affinché «le assunzioni relative alle Forze armate, in analogia a quanto stabilito nella legge n. 89 del 2005 con l'articolo 1 comma 4-*bis* per la Polizia di Stato e in ragione di equità nelle assunzioni nella pubblica amministrazione, siano effettuate in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze prioritarie» dell'amministrazione, «nonché ... la graduale incorporazione entro l'anno 2007 degli Ufficiali idonei esclusi dai concorsi citati in premessa,» o in via subordinata venga mantenuta «aperta la graduatoria, come previsto dalle leggi vigenti,» mandando al «recupero, con successive assunzioni,» gli «ufficiali che allo stato attuale risultino esclusi» dalla graduatoria. Rispetto e relativamente all'obiezione prima avanzatami da parte di alcuni colleghi, secondo i quali l'ordine del giorno G3 non sarebbe attinente alla materia del provvedimento, ricordo che anche il G1, della Commissione, interviene riguardo al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, pur non essendo lo stesso oggetto del provvedimento in esame.

il disegno di legge che stiamo per approvare è stato licenziato dalla Commissione con parere unanime. La Commissione aveva approvato, all'unanimità, un emendamento che estendeva la possibilità di derogare al divieto di autorizzare missioni

Poiché però esisteva la preoccupazione che l'approvazione di tale emendamento comportasse il riesame ovvio del decreto-legge da parte dell'altro ramo del Parlamento

materia direttamente inerente al Ministero della difesa, riguarda l'Arma dei Carabinieri che, notoriamente, ha una dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno.

Signor Presidente, onorevoli senatori, Forza Italia voterà a favore di questo provvedimento che consente di mantenere in servizio, fino al 31 dicembre 2006, un nucleo consistente di agenti ausiliari della Polizia di Stato che altrimenti verrebbe congedato proprio in questi giorni. La dispersione di 1.316 professionalità, come quelle degli agenti ausiliari che hanno frequentato il 63° e il 64° corso, è un lusso che non possiamo permetterci, soprattutto in questi ultimi tempi in cui il tema dell'ordine e della sicurezza pubblica costituisce una

e in alcune Regioni, come la Campania, che purtroppo è un triste esempio balzato al disonore della cronaca, si è trasformato in una vera e propria emergenza. questo Governo, a fronte della crescente domanda di sicurezza da parte delle nostre comunità, non ha adottato misure radicali e strutturali,

nel quale si prevedeva il trattenimento in servizio, fino al 31 ottobre 2006, degli agenti ausiliari del 63° corso. Tuttavia, agli ausiliari occorre garantire una soluzione definitiva, altrimenti si rischia di trattenerli in servizio fino al 31 dicembre 2006 ma di perderli già dal primo gennaio 2007: ciò sarebbe catastrofico sotto il profilo del controllo del territorio. In proposito, vorrei ricordare che il Governo Berlusconi ha reso effettivi quasi 11.000 ausiliari nei ruoli dell'Arma dei Carabinieri e alcune migliaia nella Polizia di Stato e nelle altre forze dell'ordine: non è una questione di numeri, ma occorre attribuire importanza, anche attraverso i numeri, al ruolo che le Forze dell'ordine rivestono. È necessario, quindi, che questo Governo manifesti un impegno chiaro nel destinare maggiori risorse finanziarie alle forze di polizia, per risolvere una volta per tutte la questione della precarietà, per garantire risorse umane, mezzi e tecnologie in grado di rispondere in maniera adeguata al bisogno di sicurezza che l'opinione pubblica richiede sempre più insistentemente. Purtroppo, non solo questo impegno ad oggi non è stato assunto, ma di contro, nella manovra finanziaria per il 2007 alcune disposizioni dimostrano il contrario: un totale, inaccettabile disimpegno. L'articolo 57 del disegno di prevede per i Corpi di Polizia la possibilità di effettuare assunzioni di personale per un contingente complessivo non superiore a 1.000 unità, senza specificare, peraltro, come tale personale venga ripartito tra i vari Corpi di Polizia. Questa cifra, ovviamente, non è sufficiente ad affrontare in modo serio il tema dei precari, né a garantire un maggior controllo sul territorio. Vorrei ancora ricordare che il Governo Berlusconi aveva previsto per l'anno 2006, con la scorsa legge finanziaria, l'assunzione di ben 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. però ancora sottolineare la gravità della soppressione contenuta nell'articolo 33 della finanziaria, delle prefetture, delle questure, dei comandi dei Vigili del fuoco nelle province con popolazioni inferiori ai 200.000 abitanti. Questa soppressione è prevista anche per le Province del Sud d'Italia ad alta densità criminale e dove la lotta alla mafia dovrebbe essere più capillare. Misure tutte che dimostrano una pericolosa insensibilità di questo Governo ai problemi della sicurezza e una scarsa attenzione al grande

per il bene dei cittadini, un'inversione di tendenza di questo Governo in tema di sicurezza, con radicali modifiche degli articoli della finanziaria e maggiori previsioni di spesa.

Gruppo voterà a favore del provvedimento in esame, che prevede il prolungamento fino al 31 dicembre 2006 del trattenimento in servizio di 1.316 agenti ausiliari della Polizia di Stato che hanno frequentato il 63° e 64° corso di agente ausiliario. Essi sono gli ultimi poliziotti entrati nella Polizia di Stato dopo la cessazione della leva obbligatoria; ne sono stati incorporati 566 il 1° aprile del 2004 e 750 il 25 ottobre del 2004, quindi, con una anzianità almeno biennale, nel corso della quale hanno potuto acquisire conoscenze, esperienze e professionalità che non possono essere sottovalutate e che non devono soprattutto essere disperse. La conversione del provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, consente di mantenere in servizio questo nucleo consistente di agenti che sarebbe stato congedato entro il corrente mese di ottobre. Gli agenti interessati a tale proroga sono impegnati in compiti operativi sul territorio, fra la gente, garantiscono una visibile presenza dello Stato, secondo l'obiettivo del Governo di mettere in atto azioni incisive per contrastare il terrorismo e la criminalità, anche attraverso il potenziamento della polizia di prossimità che, laddove è organizzata, determina una sostanziale diminuzione della criminalità e una percezione di maggiore sicurezza da parte dei cittadini. Dunque, saranno preservati per i prossimi mesi i mezzi e soprattutto gli uomini necessari alla Polizia di Stato per continuare la propria efficace azione di controllo del territorio. Bisogna considerare che il predetto personale è stato reclutato in parziale sostituzione di quello annualmente cessato dal servizio, per cui la sua eventuale mancata immissione in ruolo avrebbe come grave conseguenza la perdita di un'importante risorsa per l'amministrazione della pubblica sicurezza, che causerebbe l'inevitabile riduzione della forza effettiva della Polizia di Stato, con l'incidenza negativa sulle esigenze di servizio e sulla funzionalità dei servizi stessi, nel mentre si accrescono le necessità di intervento, come le vicende di Napoli evidenziano. Peraltro, il mancato trattenimento in servizio di questo personale configurerebbe una scelta inopportuna anche sotto il profilo di una corretta gestione delle risorse umane, perché determinerebbe perdita dell'investimento già sostenuto per la formazione di questi agenti che hanno prestato - come già ricordato - almeno due anni di servizio operativi. Il provvedimento ripropone, nella sostanza, il contenuto del decreto-legge n. 135 del 2006, convertito in legge nella fase iniziale della presente legislatura, nel quale si prevedeva il trattenimento in servizio, fino al 31 ottobre 2006, degli agenti ausiliari frequentatori del 63° corso ed onora un impegno assunto dal precedente Governo a seguito di un ordine del giorno presentato nel corso del dibattito di conversione del decreto-legge 45 del 2005, riferito alla stabilizzazione degli agenti ausiliari

al Ministro dell'interno di autorizzare il trattenimento in servizio degli agenti ausiliari frequentatori del 63° e del 64° corso che ne facciano domanda. Alla collega Casellati ricordo che l'articolo 57, comma 2, della legge finanziaria destina il 20 per cento del fondo relativo alle assunzioni alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato, innovazione non irrilevante presentata dal Governo. In conclusione, colleghi, signor Presidente, ritengo che a questo ulteriore prolungamento in servizio dovrebbe seguire un impegno del Governo a stabilizzare definitivamente questi agenti, com'è accaduto in passato per gli ausiliari

perché nel corso del 2007 sia risolta definitivamente questa situazione di precarietà, rassicurando questi giovani lavoratori e soprattutto la Polizia di Stato, che altrimenti si troverebbe in grave difficoltà nell'assolvere i normali servizi d'ordine e sicurezza pubblica. È indubbio che il problema della sicurezza necessita di un dibattito molto più approfondito, posto che esso, come ho già specificato, non può essere risolto con provvedimenti d'urgenza come questo. I recenti fatti avvenuti a Napoli confermano che la sicurezza è un problema e un bene comune, quindi è fondamentale avere delle forze dell'ordine motivate, per contrastare sia le nuove minacce del terrorismo interno ed esterno, sia i reati tipici di criminalità diffusa (scippi, rapine, furti e contraffazioni) e soprattutto quei reati che hanno consentito la creazione di grandi patrimoni illeciti derivanti dal traffico di persone, droga e armi, che insidiano la legalità e lo stato di diritto. In particolare, in questo ultimo settore, occorrono per l'attività investigativa professionalità specifiche e di alta qualità. Vorrei - e concludo - ricordare che il trattenimento in servizio di 1.316 agenti di Polizia va visto come un atto dovuto, mentre l'emendamento approvato alla Camera da noi sostenuto e ripresentato in questa sede come ordine del giorno, che concerne gli ufficiali dei Carabinieri in ferma prefissata, riguarda una questione di piccola entità, ma anch'esso aiuta le forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità organizzata. Disporre di un numero adeguato di militari già formati, con esperienza e affidabilità fuori discussione, è, dunque, utile alla causa della sicurezza ed è per queste ragioni, signor Presidente e colleghi, che il nostro voto è determinatamente favorevole favorevole a questo provvedimento.